DISEGNO DI LEGGE Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonché di finanziamento delle opere per il G8

modifiche e integrazioni che, complessivamente, hanno portato sensibili miglioramenti o, comunque, hanno tenuto

Per quanto riguarda l'articolo 1, relativo all'adeguamento dei prezzi dei materiali di costruzione,

anche alle variazioni intervenute nel campo di materiali come il legno e la plastica. La specificazione relativa deve essere fatta con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

cioè la possibilità da parte di alcuni enti mutualistici a struttura privata di poter derogare

al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. che prevede l'abrogazione della norma prevista nella legge 6 agosto 2008, n. 133, cioè lo 0,50 per cento al personale tecnico degli enti locali

la corresponsione di incentivi nella misura pari al limite della retribuzione annua (quindi è un'importante apertura al personale degli enti locali) quando le suddette attività sono sviluppate all'interno degli enti stessi. È stata introdotta un'ulteriore norma di semplificazione degli appalti cosiddetti minori; pertanto per appalti

di sforare l'anno finanziario 2008 e contengono tecnicalità che consentono di effettuare i bandi

ma al credito e agli investimenti, quindi si estende l'applicabilità della norma in quanto si crea una specie di fondo rotativo;

della legge fondamentale di liberalizzazione del settore dell'autotrasporto, si introducono, qualora si faccia ricorso a contratti scritti tra autotrasportatori e mittente, delle norme di trasparenza del contratto e quindi di moralizzazione del settore, rendendo evidenti sia sul contratto, sia sulla fattura importantissime voci di prezzo non derogabili come, ad esempio, il costo del carburante; in tal modo flessibile il contratto in ragione delle oscillazioni del costo del carburante.

della possibilità per le aziende in amministrazione straordinaria di derogare all'articolo 2112 del codice civile

chiariva che anche gli enti pubblici che avevano usufruito della possibilità di non

immediatamente successivo al terremoto potevano usufruire della restituzione graduale nella misura del 40 Non abbiamo voluto approvare emendamenti al testo in quella fase, poiché ritenevamo che tale norma fosse già contenuta nel testo del decreto emanato dal Governo. La modifica proposta dalla Camera è da un lato chiarificatrice, soprattutto perché è diretta nei confronti degli enti previdenziali che ancora avevano dubbi interpretativi, ma dall'altro lato conferma l'impostazione che aveva dato il Senato, perché, pur chiarendo che anche gli enti pubblici possono far ricorso a quelle norme di vantaggio,

*(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori del Governo, arriva oggi in Aula in terza lettura il decreto-legge

Molte sarebbero le considerazioni da fare, nel metodo e nel merito, che volutamente risparmio. Voglio evidenziare solo due aspetti su tutti.

È comunque il sintomo di sofferenze ancora deboli, ancora prive di impatti significativi, ma di già evidenti disagi che trovano risposta in provvedimenti confusi, pasticciati e indecorosi.

e riproposta o, per meglio dire, imposta dalla Lega evidentemente con maggior successo in Commissione alla Camera. La norma, ripristinando il 2 per cento dei costi sulle progettazioni fatte *in house* dagli enti locali, determina di conseguenza minori entrate per lo Stato, sottraendo così risorse preziose destinate all'ordine pubblico, alla sicurezza e alla difesa. È evidente che un provvedimento così congegnato è per noi del tutto inaccettabile soprattutto nella modalità proposta. Scusate, colleghi, ma sarebbe davvero auspicabile che le vostre beghe le risolveste a monte, senza forzare norme e *iter* procedurali con tempi assolutamente inadeguati di esame degli atti. Questo provvedimento però - questa è la seconda riflessione è anche il frutto di un altro aspetto particolarmente negativo, dovuto al combinato disposto, da un lato, di una coperta troppo corta nelle risorse, che tirate da una parte, inevitabilmente scoprono l'altra. Ma soprattutto, dall'altro lato, è il sintomo più evidente di una degenerazione della decretazione d'urgenza. Guardate che prima o poi finirà per ritorcersi anche contro voi stessi. È lo snaturamento dell'*iter* ordinario del procedimento legislativo che state perpetrando sistematicamente dall'inizio di questa legislatura, con provvedimenti a casaccio, non curanti spesso degli effetti che producono sia sul piano amministrativo con tagli o mancate idonee coperture, sia sul piano, ancora più grave, della concretezza reale delle cose. E comunque, vedendo fiduciosi che spesso le raccomandazioni garbate e gli inviti sommessi hanno più effetto degli urli e degli strepiti, torniamo ad invitarvi, come si dice in questi tempi, pacatamente e serenamente a ripristinare le prerogative proprie del Parlamento. In buona sostanza, faccia il Parlamento le riforme e le leggi necessarie al Paese. Si riporti nelle Aule e nelle Commissioni parlamentari il confronto di merito sui problemi. E non limitatevi, limitandoci, alla semplice ratifica di provvedimenti d'urgenza o a pasticciare impropriamente gli stessi. la prova provata di ciò che ho appena detto è proprio l'emendamento che il Governo, impropriamente ed ostinatamente, aveva proposto ed imposto proprio qui al Senato, sulla storia infinita di Alitalia, emendamento che introduceva ulteriori deroghe e sospensive alla legge Marzano già in precedenza abbondantemente rivisitata e che peraltro la estendeva pericolosamente, in termini assolutamente generici, e di conseguenza applicabile ad ogni futura necessità, determinando nel breve periodo un possibile sfondamento degli equilibri di bilancio, come vi avevamo segnalato molto garbatamente. Lo stesso emendamento dallo stesso Governo alla Camera è stato ritirato. Il Governo ha così effettuato di fatto un ravvedimento operoso, che apprezziamo ma che era assolutamente evitabile se solo avesse, e aveste, dato semplice ascolto alle nostre garbate raccomandazioni. Confidiamo per voi, ma soprattutto per il Paese, che vi assicuriamo teniamo in particolare considerazione, che per le prossime volte possiate darci maggiore ascolto. Altri colleghi interverranno per presentare emendamenti con i quali ci ostiniamo a dare l'ulteriore nostro contributo al miglioramento di un provvedimento che giudichiamo davvero saccheggiato e pasticciato. Mi voglio permettere un'ultima riflessione conclusiva riguardante l'autotrasporto. Una riflessione che, colleghi della maggioranza, vuole essere anche sommessamente un monito per il futuro. Attenzione, il mondo dell'autotrasporto è un settore da maneggiare con cura in ragione di due aspetti essenziali: il primo, derivante dalla consapevolezza delle condizioni di lavoro, spesso infami a cui sono sottoposti autisti e padroncini a causa di una persistente deregolamentazione in termini di concorrenza e di norme di reciprocità adeguata agli altri Paesi membri dell'Unione europea e soprattutto di una non adeguata azione di controlli, che costituisce peraltro un terribile fattore di insicurezza sulle nostre strade. Il secondo, derivante invece dalla consapevolezza della fragilità del nostro sistema Paese che, anche in ragione di quanto avvenuto proprio lo scorso anno di questi tempi, rischia di consegnarsi prigioniero, di un settore che nel tempo ha costituito per il commercio non solo la naturale forma di approvvigionamento e di distribuzione di merci e di derrate, ma anche impropriamente, direttamente o indirettamente, il settore di stoccaggio delle merci. Guardate - e concludo - questo è il sintomo più evidente di un Paese che non riesce a fare della logistica e dell'integrazione modale dei trasporti il proprio punto di forza e che rischia di pagare un prezzo troppo alto, direi perfino insopportabile, sul piano dei costi e della concorrenza.

Un forte salto di qualità nell'efficienza delle infrastrutture e dei trasporti rappresenta uno dei passaggi essenziali per restituire competitività al nostro sistema produttivo e per mettere in rete, nell'ambito del mercato europeo e globale, il nostro sistema Paese. Il nostro Paese, anche a causa della modalità con cui negli anni Novanta ha proceduto alla politica delle privatizzazioni e dopo la delocalizzazione produttiva verso l'Est europeo e asiatico, ha dimezzato la sua capacità di crescita rispetto alla media europea. L'inserimento strutturale della grande rete di trasporto europeo e mondiale potrà dare all'Italia un contributo aggiuntivo decisivo ad una maggiore crescita economica. Sappiamo che nel nostro Paese il trasporto delle merci è assicurato per l'80 per cento dal vettore stradale, che subisce quindi i condizionamenti della congestione del traffico, con riflessi negativi sulla sicurezza della circolazione, oltre che gli alti costi dei carburanti e le difficoltà connesse ai rapporti contrattuali con la committenza. Con questo decreto si intende riconoscere il maggiore costo sopportato dall'autotrasporto per il gasolio nei primi mesi del 2008 e negli ultimi del 2007, ad integrazione degli altri provvedimenti deliberati negli ultimi mesi, che hanno inteso anche - lo voglio ricordare al senatore Filippi - dare attuazione agli impegni assunti dal precedente Governo allorché ha dovuto fronteggiare il blocco dei TIR, che, lo scorso dicembre, causò una perdita di produzione di circa 3 miliardi di euro. Va sottolineato che, per la prima volta, le misure economiche favoriscono la strutturazione delle imprese, gli investimenti in logistica e l'accesso al credito delle aziende del settore. Sul piano normativo il provvedimento chiarisce e rende applicabili le nuove norme introdotte dalla legge n. sui rapporti contrattuali tra vettori e committenti, allo scopo di incentivare i contratti scritti, penalizzare quelli verbali e favorire così fenomeni di emersione. Possiamo dire che il punto di riferimento più qualificante di questa norma è la crescita della qualità del servizio fornito dagli autotrasportatori, che vedono riconosciuto il loro ruolo fondamentale nell'economia del Paese. Questo provvedimento, insieme all'approvazione definitiva, dopo il dibattito parlamentare, nel prossimo Consiglio dei ministri, del decreto legislativo che introduce correttivi alla riforma del 2005, qualifica bene l'impegno del Governo nei confronti dell'autotrasporto. Per questo Governo è motivo di particolare soddisfazione l'aver evitato al Paese un nuovo fermo dei TIR, che avrebbe avuto conseguenze disastrose nella già difficile congiuntura economica. In conclusione, vorrei dire al senatore Filippi che questo Governo riprenderà il piano della logistica approvato all'inizio del 2006

«La 1a Commissione permanente, esaminate le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. Esaminati i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo». parere non ostativo». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta». parere di nulla osta». «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

pubblici alle fondazioni o agli enti privati. Oggi essa viene ancora una volta estesa anche agli enti previdenziali, agli autonomi e ai professionisti. Ebbene, vorrei ricordare a quest'Aula di cosa stiamo parlando: in sostanza, non si applica la

1.103 e 1.104, l'articolo prevede l'affidamento dei lavori con procedura negoziata, senza pubblicazione di bando di gara, con inviti rivolti ad almeno cinque soggetti, per importi che vanno da 100.000 a 500.000 euro. Questo è un problema che si può riscontrare soprattutto negli enti locali, dove molto spesso le gare vengono «spacchettate» e i 500.000 euro, in varie gare, possono diventare

Il relatore ha riferito che la Camera ha introdotto la norma finalizzata a rielevare l'incentivo ai dipendenti pubblici, al personale tecnico degli enti locali in particolare, dallo 0,5 per cento che era stato determinato con il decreto-legge n. pur in un contesto di limitazioni nella possibilità di erogazione di questi incentivi. Senonché il relatore non ha riferito che questa disposizione, che ovviamente comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, viene viene coperta con l'abrogazione del comma 8 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112. PRESIDENTE. Le chiedo scusa, collega Legnini. Senatore Cicolani, il collega Legnini si sta rivolgendo a lei direttamente.

per cento della misura di questo incentivo. Senonché, il comma 8 era collegato al comma 17 dell'articolo 61, il quale istituiva un fondo, alimentato dall'economia di spesa

inclusa l'assunzione di personale in deroga alle restrittive norme vigenti e, inoltre, al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, incluse le forze dell'ordine, le agenzie fiscali, gli enti di ricerca, le università

precedentemente stabilita dei 200 milioni di euro dal decreto-legge n. 112. Tradotto: con questa disposizione, con la quale si ripristina - seppure parzialmente - la possibilità (secondo noi nel merito correttamente, perché ritenevamo quella norma errata) di erogare al personale tecnico degli enti locali l'incentivo per la progettazione fino al 2 cento, togliete i fondi alla sicurezza pubblica e al personale del comparto della sicurezza. È un vero e proprio pasticcio, signor Presidente, che mi auguro il Governo voglia

considerazioni: la corsa forsennata alla quale abbiamo partecipato - ahinoi - in questi mesi a convertire i decreti sta determinando un vero e proprio caos normativo, con errori di vario genere e necessità di continui ripensamenti e interventi correttivi; e questo è uno di quelli.

diverso, a partire dalla conversione del decreto-legge n. 185, oggi all'esame della Camera e che mi auguro non venga qui blindato. seconda considerazione è rivolta alla maggioranza e al Governo: per favore, nel momento in cui continuate a togliere fondi per la sicurezza, non parlate più delle vostre buone intenzioni sulla sicurezza. Ogni atto contraddice i propositi che voi Se volete recuperare su questo terreno un minimo di dignità e di coerenza tra ciò che si dice e ciò che si fa, accogliete uno di questi due emendamenti, per ripristinare quel minimo di fondi per la sicurezza pubblica che era stato previsto con il decreto-legge n. 112 a fronte di tagli che furono all'epoca corposi. Lo ricordo: si trattava 800 milioni di euro in meno per il comparto della sicurezza, che furono in minima parte compensati con quel fondo che oggi viene sostanzialmente svuotato per dare più fondi - che erano stati erroneamente tolti - al personale tecnico dei Comuni e delle Province.

la maggioranza, non il Governo - ha riconosciuto la fondatezza della nostra obiezione, che non riguarda il che non riguarda il tema della copertura finanziaria in senso tecnico. È chiaro che la Commissione bilancio non poteva e non doveva effettuare rilievi

di pasticci compiuti con ordini del giorno, raccomandazioni: è una soluzione che non ci soddisfa. Noi insistiamo per la votazione di questi emendamenti e ciascuno si assuma la propria responsabilità: state nuovamente togliendo fondi ai Carabinieri, alla Polizia, al comparto della sicurezza e predicate l'esatto contrario un giorno sì e l'altro pure. Signora Presidente, vorrei puntualizzare un aspetto al senatore Legnini per evitare che questa sera si ingeneri un elemento di confusione attorno ad una decisione che il Governo e la maggioranza intendono assumere in maniera trasparente. Ha ragione il senatore Legnini a porre, come ha fatto, la questione presentando due emendamenti.

trovare una soluzione che risolva questo problema, il che significa non incidere sugli stanziamenti precedentemente disposti e presentare un ordine del giorno.

il ripristino della situazione *ex ante*, quindi l'eliminazione di quanto disposto da tutti i Gruppi alla Camera, oppure l'individuazione di una diversa copertura per questo emendamento che originariamente tutti avevamo valutato positivamente, dato che nel testo originario la

**Il Senato non approva.**

considerata l'introduzione normativa operata con il comma 10-*quater* dell'articolo 1 del provvedimento in esame, impegna il Governo a considerare il ripristino delle risorse originariamente indirizzate alle Forze dell'ordine, alla giustizia ed alla contrattazione integrativa.

all'interno del decreto anticrisi. C'è però anche da dire che nella discussione della finanziaria, in cui abbiamo riproposto lo stesso problema, con in più una richiesta di finanziamento per il 2009,

Signora Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte ad un nuovo decreto-legge - sarebbe forse il caso di chiamarlo decreto *omnibus* - varato dal Governo per far fronte alle ennesime questioni chiamate urgenti e necessarie. È un testo che giunge al voto finale in Aula immacolato, senza che le Commissioni competenti abbiano potuto apportare alcuna modifica, per le richiamate ragioni di necessità ed urgenza. Ritorna ancora una volta di attualità la questione, che abbiamo sembra lamentato, del continuo ricorso alla decretazione d'urgenza per affrontare problematiche non omogenee quindi in contrasto con le disposizioni e la giurisprudenza che regolano l'uso del decreto-legge. Sia ben inteso: noi consideriamo gli obiettivi perseguiti dal decreto-legge meritevoli e di grande importanza, ma avremmo preferito discuterli, come penso avrebbero preferito anche i parlamentari della maggioranza, approfondirli e magari, anche con il nostro contributo, migliorarne la portata. Grazie, signora Presidente.

Non si può certo essere contrari (e noi sottolineiamo di essere a favore degli obiettivi perseguiti) a norme che cercano di sollevare e dare respiro dalla drammaticità in cui vivono oggi alcuni settori vitali del nostro sistema produttivo. Pensiamo alle infrastrutture, la cui realizzazione va certamente portata avanti non solo in termini di viabilità ed esigenze del Paese ma anche in termini economici. Pensiamo ai settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, che già subiscono, nei gravi costi, le bizzarrie del petrolio oppure la concorrenza sleale di chi spesso arriva da Paesi esteri. Sulla questione del petrolio, annuncio che il nostro Gruppo presenterà un'interpellanza urgente al Ministro, perché non è giustificabile che i costi del petrolio siano caduti, in pochi mesi, da 146 dollari al barile a circa 40 (cioè di due terzi), mentre i prezzi

conseguenti agli eventi sismici che colpirono nel 1997 alcuni Comuni delle Regioni Umbria e Marche e prevede interventi in materia di protezione civile, con particolare riferimento al grande evento della presidenza italiana del G8. È un evento importante, al quale teniamo, ma certamente si doveva guardare, per questa soluzione, da altre parti.

Con il solito colpo di genio, si affrontano questioni sicuramente importanti ma si continua con i soliti "giochetti" (come lamentano soprattutto i nostri colleghi del Sud appartenenti al nostro Gruppo UDC, SVP e Autonomie) a danno delle aree più critiche del nostro Paese. Mi riferisco all'impiego delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate che, in questo decreto-legge, vengono utilizzate per interventi non riconducibili alle finalità del Fondo medesimo. Al di là della violazione delle finalità, quello che occorre evidenziare è che questa tendenza, o meglio questa cattiva abitudine, rischia di pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a carico delle medesime risorse del Fondo, considerato anche che le risorse del FAS sono prioritariamente destinate ad integrare le risorse comunitarie e non possono risultare di ammontare inferiore a quello concordato in sede europea. Inoltre (anche qui sottolineiamo la giusta lamentela dei colleghi che rappresentano il Meridione d'Italia), il tutto consta nello scippo di circa 1,3 miliardi di euro dalle somme da destinare al Mezzogiorno: siamo ai limiti del sostenibile. Tornando al contenuto del provvedimento, ci chiediamo se nell'approntare gli interventi contenuti nell'articolo 2, riguardante il recupero della competitività di alcuni nostri settori colpiti dall'impennata dei prezzi dei prodotti petroliferi, perché non siano state previste misure strutturali e permanenti per favorire i settori individuati: l'agricoltura, la pesca professionale e l'autotrasporto, che meritano interventi seri e concreti, strutturali e non piccole, anche se condivisibili, misure tampone, al fine di evitare che, terminato l'"effetto decreto", i settori in causa tornino a lamentare le stesse lacune in termini di competitività. Proprio sul prezzo del petrolio, insisto: sarebbe una prima misura urgente per il settore dell'autotrasporto. Inoltre, vorrei soffermarmi sulla strana vicenda della norma recata dall'articolo 3-*bis*, che un emendamento del relatore alla Questa disposizione vedeva disapplicata la norma civilistica in materia di diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda; si trattava di una norma diretta ad evitare che nella vicenda Alitalia potessero subentrare ulteriori problemi nel passaggio di lavoratori licenziati dalla vecchia alla nuova compagnia. Si era tentato, cioè, di sacrificare sull'altare dell'Alitalia un'altra volta anche i diritti di tutti quei lavoratori di grandi imprese in crisi. Pensavamo ad un rinsavimento dello Stato quando c'è stata questa soppressione ma ci siamo dovuti ricredere nel momento in cui abbiamo ritrovato la stessa norma nel decreto anticrisi, più precisamente all'articolo 14, e ci chiediamo allora quale sia la *ratio* di questo giochetto di «leva qui e metti là». Vorrei dire che noi siamo sempre stati in una posizione di assoluta lealtà - lo diciamo al Governo - e di contribuzione al processo e percorso di costituzione dei provvedimenti; ci siamo resi disponibili a svolgere un'opposizione costruttiva (lo abbiamo anche sottolineato in dichiarazione di voto sulla fiducia) solo nell'interesse del Paese e ci siamo sempre augurati di trovare momenti di condivisione: ma il Governo appare sottrarsi sempre di più al confronto parlamentare. La convulsione dei momenti che stiamo vivendo, la crisi che stiamo toccando con mano, ogni giorno sempre di più, ci dimostra che non è probabilmente questa la strada migliore per procedere nell'interesse generale. C'è l'offerta di collaborare per risolvere una grave crisi che grava su tutte le nostre famiglie e su tutti i nostri operatori economici. Il Governo è veramente chiamato a cercare cercare e a chiedere la collaborazione di tutti, che noi abbiamo sempre offerto. Non c'è un disegno organico e una visione strategica per affrontare questa crisi: lo dimostra ulteriormente il decreto che stiamo discutendo. Chiediamo al Governo e, in particolar modo, alle politiche economiche dello stesso di affrontare la situazione con una visione strategica, di cui vi sia chiarezza in quest'Aula affinché questa chiarezza venga trasmessa al Paese, dando con questo anche un senso di maggiore sicurezza: esattamente quello che ha chiesto il Presidente del Consiglio, che però nei fatti non si rispecchia in quest'Aula. Ci viene chiesto di avere ottimismo sulle vicende che riguardano il Paese: dobbiamo essere noi per primi, il Parlamento, ma penso anche il Governo, a trasmettere questa tranquillità. In conclusione, questi sono tutti elementi che ci portano a considerare gli obiettivi del provvedimento in esame molto importanti; ma il provvedimento stesso incongruo alla portata delle iniziative che invece dovevano essere previste, non del tutto soddisfacente nel metodo e in particolare inopportuno e assolutamente errato per la copertura finanziaria che tocca in larga parte le speranze e le ragioni dei cittadini del Mezzogiorno del nostro Paese.

poco fa. Reputiamo che alla Camera ci sia stato un peggioramento - lo dico al relatore - relativamente agli appalti a trattativa privata. È assurdo: si può avere anche un provvedimento anticrisi, provvisorio, di un anno o due, ma portare la trattativa privata di norma, su 3 miliardi di euro all'anno che spendono le amministrazioni pubbliche, a 500.000 euro mi sembra veramente esagerato e a danno totale della trasparenza. Credo che sia importante rilevare questo. Spero che il Governo

l'idea di un quadro completo sia di una politica economica che di una politica verso la Protezione civile.

derogare a una sentenza della Corte costituzionale solo per una Regione. Credo sia uno schiaffo alla dignità delle persone e al diritto perché la Corte costituzionale ha detto che tutti i dipendenti pubblici e i datori di lavoro di tutta Italia dal 1992 a oggi non hanno diritto nel bene e nel male all'esenzione. Oggi dite: è solo per una Regione o una Regione e mezzo. Credo che sia sbagliato; potevate qualificarvi dicendo che da oggi in poi quella sentenza si applica a chi ha beneficiato della sospensione dal 1992. Ci sono 22 posti in Italia in cui si è attivata questa sospensione, ad iniziare dal Piemonte. C'è dentro perfino Arcore

allo sfizio di qualcuno, al beneplacito di un Ministro o di un Presidente del Consiglio in carica. Di fronte alle calamità naturali credo che un diritto lo debba fissare in maniera assoluta la legge perché chi chi ha avuto una disgrazia del genere è ancora più debole di chi entra nel tunnel delle malattie. Ecco perché - ripeto - il nostro voto, sollecitandovi a provvedere anche per il Molise, è di astensione. Signora Presidente, onorevoli colleghi senatori, gentili membri del Governo, sono qui oggi a ribadire il voto favorevole della Lega Nord alla conversione di questo decreto, come già ho fatto a nome del mio Gruppo in prima lettura lo scorso 20 novembre. Il decreto ritorna da noi al Senato dopo che la Camera dei deputati ha operato alcune modifiche. Vorrei sottolineare come grazie a due emendamenti delle Lega Nord, che sono stati fatti propri dalla Commissione ambiente e sono stati elaborati in collaborazione con il Ministero, si siano fatti due passi importanti nella direzione di fornire ai sindaci strumenti fondamentali che permettono ai Comuni - soprattutto a quelli piccoli di realizzare le loro opere pubbliche in un modo che sia più economico e con procedure, quando possibile, più rapide. Stiamo parlando - è stato evocato varie volte dagli interventi che mi hanno preceduto - del ripristino dell'incentivazione del 2 per cento a base di gara per le progettazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche e dell'importo dei lavori per i quali è ammessa la trattativa privata.

che permetterà la valorizzazione delle risorse interne ai nostri enti locali nell'ottica del buon governo e del risparmio delle risorse pubbliche, senza creare alcun elemento di conflittualità o di concorrenza con il mondo imprenditoriale privato. Non c'è bisogno che stia qui a fare i conti. Mi fa piacere che anche il senatore Legnini che mi ha preceduto, concordi sul merito del

Abbiamo poi parlato dell'altro punto importante, ossia l'innalzamento da 100.000 euro a 500.000 euro dell'importo per i lavori ammessi alla trattativa privata,

sono nell'ottica di uno snellimento e di un'economicità delle opere realizzate dagli enti locali. Su tale aspetto penso che non ci sia nessuno che possa dire il contrario da qualunque parte di quest'Aula.

Non c'è stata assolutamente alcuna pressione. Noi siamo una forza di Governo e insieme agli alleati lavoriamo e operiamo per governare al meglio questo Paese. Oltretutto, ritengo che non sia affatto vero che vengano tolte risorse alla sicurezza. Se così fosse, noi saremmo i primi ad opporci a una simile soluzione.

modifiche agli importi destinati alla sicurezza; anzi, noi e tutta la maggioranza ci batteremo ed opereremo sempre perché le

Signora Presidente, onorevoli colleghi, nella rilettura del disegno di legge n. 1152 troviamo nuovamente punti di non condivisione, come vediamo che alcuni emendamenti da noi sostenuti in prima lettura e respinti dall'Assemblea sono stati invece ripresi dalla Camera e approvati. Vorrei partire dall'articolo 1. Ci imbattiamo nuovamente nella non applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici per associazioni e fondazioni. Ma questa volta la non applicazione viene estesa a soggetti che svolgono tutela previdenziale obbligatoria degli ordini professionali. Come si può pensare che enti di gestione che hanno migliaia di iscritti non applicano la trasparenza quando hanno necessità di forniture di servizi ed appalti?

Il risparmio, come ha detto il senatore Legnini, avuto dalla finanziaria era stato messo in un fondo del bilancio che andava a finanziare voci della sicurezza pubblica. Ora quel fondo non c'è più. La sicurezza ancora una volta è stata solo uno slogan elettorale. Ma il primo capitolo ad essere tagliato, quando servono risorse, è quello Viene introdotto il concetto che per velocizzare alcuni piccoli appalti per gli importi che vanno da 100.000 a 500.000 euro (parliamo

Riteniamo prima di tutto che non si può intervenire sul codice appalti - vorrei richiamare sull'argomento sia il presidente Grillo sia il senatore Cicolani modificando parti isolate e non facendo un progetto complessivo. Abbiamo lavorato a luglio insieme in Commissione sul codice. Oggi ci troviamo di fronte ad interventi *spot* e non organici. Nel particolare, la pericolosità di vedere reiterare più volte su stessi appalti in più *tranche* le stesse imprese in modo tale che non superino la somma di 500.000 euro è una realtà. Anche qui, questo Senato deve rendersi conto che il Paese ci ascolta e noi stiamo dicendo che è possibile eludere la legge e fare appalti a trattativa diretta per importi superiori a 500.000 euro. Rileviamo con gran soddisfazione che l'articolo 3-*bis* del decreto, in cui era prevista la non applicazione dell'articolo 2112 del codice civile è stato soppresso. Era un fatto gravissimo che avevamo sottolineato al Senato. Come si può o come si poteva pensare che le operazioni previste da un commissario straordinario del programma di salvataggio delle imprese in stato di insolvenza non costituisca trasferimento d'azienda? Oggi, nella drammatica situazione economica in cui ci troviamo, le aziende avrebbero lasciato i lavoratori senza tutela

Potremmo sempre dire: «L'avevamo detto». La Camera lo ha cambiato. Ancora una volta ci sembra che si voglia migliorare l'efficienza dello Stato e in questo modo nascondere la vera realtà: togliere controlli e trasparenza. Soprattutto la competitività delle imprese fornitrici del pubblico viene meno.

che non vi sia un rapporto dialettico. Credo che la fretta tolga al Senato intero la sua capacità di confronto, la sua capacità di poter esprimere la volontà di maggioranza e opposizione anche nel creare condizioni di sinergia. Per questi motivi, il Gruppo del PD esprime voto contrario al provvedimento. Signora Presidente, il Gruppo del PdL voterà a favore di questo provvedimento, non solo perché in prima lettura lo abbiamo sostenuto convintamente ma perché riteniamo che il passaggio alla Camera abbia contribuito a migliorare il testo originale. Motivo questa affermazione riprendendo alcune critiche che i colleghi della minoranza hanno voluto rappresentare quest'oggi in Aula. Il collega Filippi, ad esempio, ha lamentato il fatto che in questa dialettica che c'è stata in Parlamento, quest'ultimo, alla fine, ha subito

siamo alla terza lettura. Nell'8a Commissione abbiamo avuto tempo e modo di approfondire vari argomenti. Abbiamo fatto anche poderose audizioni. Abbiamo ascoltato l'ANCE, l'AGI, l'IGI su un tema che oggi non è rimbalzato all'attenzione dei nostri lavori e che poi è stato all'origine del decreto d'urgenza emanato dal Governo relativo all'adeguamento prezzi per andare incontro alle esigenze delle aziende colpite da un aumento dei prezzi che aveva messo in discussione gli equilibri economici e finanziari delle stesse imprese. Quindi, credo che il Parlamento abbia fatto la propria parte. Voglio ora sottolineare gli aspetti che, a nostro modo di vedere, nel passaggio alla Camera

a predisporre il codice degli appalti del nostro Paese. Siamo l'unico Paese in Europa che nel 2006, cancellando ben 53 leggi esistenti, si è dotato di un codice che ha avuto largo consenso nell'opinione pubblica e tra gli operatori.

quel codice non dovrebbe essere mutilato ad ogni occasione con provvedimenti saltuari che nascono all'interno di norme, decreti ed iniziative. Su questo siamo d'accordo, perché quel codice,

Non mi sembra che valga organizzare una polemica sul fatto che tali enti possano procedere senza rispettare pedissequamente ed in maniera vincolistica le norme dettate dal codice perché non sono enti pubblici. Per questi enti vale certamente il carattere pubblicistico dell'attività principale, ma gli strumenti, le modalità di operare, il fatto di introdurre nei circuiti risorse cospicue che questi enti hanno, per quale motivo la loro attività adoperando le norme statutarie? Vede, collega Ranucci, non è vero che gli enti privatizzati, l'ENPAM e tutti gli altri enti che abbiamo indicato in questa norma, non operano secondo i criteri di trasparenza e di pubblicità: questi enti la trasparenza e la pubblicità la praticavano addirittura prima del codice, nel rispetto di quanto prevedeva la legge n. 109 del 1994, la famosa legge Merloni, tanto che avevano adeguato i loro statuti al rispetto di quelle norme. Il problema è di non mettere questi enti nelle condizioni di subire, ad esempio, le procedure di sospensiva del TAR essendo, appunto, enti privati, perché lo Stato nei confronti di questi enti non ha mai fornito finanziamenti o contributi. Questa estrapolazione, quindi, a parer mio è assolutamente non solo condivisibile ma comprensibile in una logica, anche se non troppo importante, di manovra anticiclica.

un segno di manovra anticiclica, nel senso che consente di fare più appalti, di farli più speditamente e di non dover aspettare due anni prima che sia concluso un appalto pubblico, con tutti i ricorsi, le valutazioni dell'offerta anomala, i rimpalli, i confronti e i dibattiti a cui purtroppo la normativa

per sveltire la realizzazione delle opere strategiche, così come - mi pare altrettanto importante tra gli aspetti qualificanti e qui non è stato ancora detto - ciò che è stato previsto in tema di autotrasporto. previsto in tema di autotrasporto. Credo che i colleghi non possano non considerare che proprio l'approvazione di queste norme, l'aver introdotto norme contrattuali che migliorano, ad esempio, la sicurezza, ha evitato il blocco dei TIR

che il provvedimento debba essere approvato. Pur con i limiti che abbiamo individuato e nei confronti dei quali abbiamo disposto la presentazione di un ordine del giorno per porre rimedio all'emendamento all'articolo 1,

***Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA

perché non riesco a sentire il senatore Legnini.

annunciato questa scansione dei lavori, volevo che fosse precisato

ci eravamo resi conto che c'era un serio problema di copertura; pertanto, avevamo convenuto che era possibile procedere alla discussione generale, ma non alla votazione

il disegno di legge autorizza il Presidente della Repubblica ad aderire al Trattato che è stato concluso nel maggio del 2005 tra Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi, Germania, Francia e Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in modo particolare per contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. Il Trattato prende il nome da Prum, la città tedesca in cui fu siglato Giova ricordare, in proposito, che la mancata sottoscrizione iniziale dell'Italia al Trattato è stata determinata solo della circostanza per cui non era previsto nel nostro ordinamento interno un sistema di gestione di una banca dati del DNA. Infatti, nel corso del 2007, il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, aveva approvato una risoluzione che impegnava il Governo a prendere le opportune iniziative volte a ratificare il Trattato di Prum e ad intervenire sulla normativa nazionale in materia. Inoltre, possiamo dire che fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 del Trattato, quando agenti di una parte contraente operano nel territorio nazionale, lo Stato italiano può provvedere al risarcimento dei danni causati dal personale straniero limitatamente a a quelli derivanti dallo svolgimento delle attività svolte conformemente al Trattato.

Ricordavo che il Trattato di Prum prevede l'istituzione di tre banche dati nazionali: la banca dati del DNA, la banca dati delle impronte digitali e il registro di immatricolazione dei veicoli. Un elemento di novità delle disposizioni del Trattato riguarda ciò che disciplina i cosiddetti *sky marshals*, ossia le scorte armate imbarcate sui voli con funzione di prevenzione degli atti terroristici e, più in generale, di prevenzione di quelle condotte che possono mettere in pericolo la sicurezza del volo. Si prevede inoltre che le parti contraenti possano istituire, al fine del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica e per prevenire i reati, pattuglie comuni o altre forme di intervento comune, nell'ambito delle quali funzionari o altri agenti di autorità pubblica partecipano ad interventi sul territorio di un'altra parte. La particolarità delle pattuglie comuni è data dalla loro finalità che non è quella di investigare su un reato già commesso bensì quella di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica e prevenire la commissione di reati. Si stabilisce, inoltre, che in situazioni d'urgenza i funzionari di una parte contraente possano attraversare, senza previa autorizzazione dell'altra parte contraente, la frontiera comune con lo scopo di adottare, in zona di confine dell'altra parte contraente e nel rispetto del diritto nazionale di questa, delle misure provvisorie e necessarie ad allontanare ogni attuale pericolo per la vita e l'integrità fisica delle persone. Concludendo, possiamo dire che il Ministro dell'interno deve informare annualmente il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione: sullo stato di attuazione delle previsioni del Trattato, sulle azioni intraprese e sugli accordi conclusi, con specifico riferimento a quelli attuativi di cui all'articolo 44 del Trattato. Infine si prevede che l'attuazione delle norme di cui al disegno

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Galperti. Ne svolgerò alcune brevi considerazioni rispetto alla relazione che ha già tracciato il senatore Divina che mi sembra abbia riportato e reso ben

sottolineandola e valorizzandola, la possibilità di realizzare un maggiore e più efficace scambio di informazioni tra i Paesi che hanno aderito e che sottoscrivono il Trattato. Così come rende agevole, quindi utile,

il lavoro presentato attraverso un disegno di legge dai senatori del Partito Democratico Rutelli e Zanda che credo abbiano fornito un contributo oggettivamente importante e abbiano consentito con il loro testo con il loro testo di arricchire, sottolineare, aggiungere alcuni istituti e alcune condizioni utili alla realizzazione delle finalità che il Trattato prefigura

il confronto all'interno del Senato guarda alla sostanza dei problemi ed è in grado di porre in atto e in essere alcune soluzioni efficaci.

dopo la discussione a votare un provvedimento importante e complesso che va nella direzione giusta rispetto a grandi questioni che tutti conoscono e che sono continuamente

principalmente per assolvere a quello che ritengo un obbligo morale. Nell'agosto 2006 ebbi l'incarico, da Sottosegretario, di coordinare il gruppo di lavoro che iniziò ad elaborare questo disegno di legge; quindi, ebbi modo di apprezzare il livello eccezionale ed eccellente della nostra Polizia scientifica e del RIS, così come apprezzammo in quella sede il lavoro della Polizia penitenziaria. Abbiamo delle polizie di eccellenza, invidiate dagli altri Paesi del mondo,

per arrivare all'elaborazione di questo disegno di legge è un discorso antico. Vorrei ricordare

rientri tra gli obblighi morali anche quello di ricordare l'enorme lavoro svolto dal compianto presidente Gianfranco Manzo, capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, che si impegnò perché potesse arrivare a conclusione questo percorso, anche utilizzando i lavori del Comitato nazionale per la biosicurezza.

e che era composto dagli organismi di polizia scientifica dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, oltre che dai componenti dell'Ufficio legislativo del Ministero.

relazione al disegno di legge che porta il mio nome come primo firmatario, ma che è quello presentato dal Governo nella scorsa legislatura. È stata ripetuta in questa legislatura una procedura, ma era talmente buono il lavoro fatto, che il disegno di legge n. 905 del Governo ha ricalcato, ha ricalcato, anche nelle virgole della relazione, il disegno di legge originario n. 1877. È un grossissimo risultato che ha visto la Commissione giustizia e la Commissione esteri lavorare in perfetta sintonia, nel senso che si era totalmente d'accordo sull'esigenza di dotare anche il nostro Paese di questo strumento di notevolissima importanza per la lotta al crimine. Si pensi soltanto al fatto che i profili del DNA estratti dai reperti rinvenuti sul luogo di un crimine commesso da ignoti muoiono nei singoli fascicoli e non vengono,

tra il reato rimasto ad opera di ignoti e la persona che viene arrestata per un altro reato. Ovviamente tutto ciò nel rispetto delle norme estremamente rigide che il Comitato nazionale per la biosicurezza ha imposto, oltre che del rispetto delle norme sulla *privacy*. Trattandosi di profili tracciati, l'accesso al nominativo riferibile a quel profilo estratto avverrebbe in un secondo momento, quando vi è sovrapponibilità dei risultati.

transfrontaliera di disporre di uno strumento di aggressione e di contrasto particolarmente efficace. Quindi, con soddisfazione, vedo l'approdo

la possibilità di uno scambio dei dati dattiloscopici, gli archivi delle impronte digitali, ad uno scambio di informazioni per prevenire reati terroristici. Determina anche la possibilità di prevedere guardie armate a bordo di aeromobili e misure incisive nella lotta all'immigrazione illegale, con

Prevede poi misure importanti nel sostegno reciproco dei Paesi per l'allontanamento degli immigrati clandestini (con misure comuni di espulsione, per via aerea, degli immigrati clandestini e con misure di allontanamento); forme di cooperazione incisive tra le forze di polizia e per un'assistenza reciproca nella verifica dei titoli di soggiorno, nelle verifiche di identità, in quelle riguardanti i luoghi di soggiorno e di residenza

nell'ottobre 2007, che però poi rimase lettera morta. Altri Paesi europei si sono mossi più celermente di noi e hanno oggi la possibilità di identificare un maggior numero di autori del reato. L'adesione a questo Trattato ci consente, finalmente, di istituire la banca dati nazionale del DNA, che verrà collocata all'interno del Ministero dell'interno, e di realizzare il laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA presso il Ministero della Giustizia, specificatamente presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia. Tutto ciò avverrà mantenendo un altissimo livello di garanzie proprio per evitare abusi o l'uso distorto delle informazioni. Con l'istituzione di questa banca dati del DNA aumenteremo significativamente l'identificazione degli autori dei reati, che oggi troppo spesso restano ignoti, e inoltre rafforzeremo la possibilità di rintracciare persone scomparse. Forse, anche al tema delle persone scomparse occorrerebbe dedicare maggiore attenzione.

volte della percentuale d'identificazione degli autori dei reati. Per fornire un solo dato, che può servire per capire l'importanza di questa banca dati nazionale del DNA, nel 2005 nel nostro Paese sono stati denunciati

l'attuale maggioranza sta portando a compimento. L'adesione a questo trattato, tra l'altro, costituisce una condizione fondamentale per la realizzazione del secondo pilastro delle politiche di sicurezza dell'Unione europea in materia di cooperazione giudiziaria e di polizia. Attraverso l'istituzione di questo casellario centrale dei profili del DNA riusciamo, evidentemente, a porre una pietra miliare fondamentale sulla struttura investigativa, soprattutto per tutta una serie di reati che trovano la loro matrice nell'identità ematica. Credo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che finalmente il nostro Paese si ponga al riparo da tutte le critiche che erano venute anche a livello internazionale sull'incapacità di aderire al Trattato di Prum (ricordo io stesso alcune che furono elevate da alcuni Ministri dell'interno alcuni anni fa sul ritardo con cui l'Italia aderiva a questo Trattato), ma soprattutto ci ponga nella condizione di far sì che gli apparati investigativi dell'Unione europea possano cooperare con il nostro Paese nelle investigazioni giudiziarie più pericolose, fra cui non possiamo dimenticare il contrasto al terrorismo internazionale. Credo che nel lavoro che è stato fatto dai colleghi che si sono occupati di questo provvedimento (in particolare desidero ringraziare il sottosegretario Alfredo Mantovano e i due relatori Mugnai e Divina), sia stato trovato un perfetto equilibrio tra le esigenze di tutela dei diritti di *habeas corpus* ed il fondamentale divieto dei trattamenti sanitari obbligatori; pertanto il prelievo delle sostanze che consentono l'accertamento del profilo del DNA rientra perfettamente nei canoni di civiltà e soprattutto di tutela della dignità umana, anche di persone che hanno commesso reati, o a cui si attribuiscono ipotesi di reato. Credo non si debba neppure sottacere il contributo che è stato portato a questo provvedimento da parte dei colleghi dell'opposizione. L'Italia si incammina insieme a tutti gli altri Paesi, quindi, verso un traguardo fondamentale nel contrasto a tutta una serie di fenomeni criminosi. Ricordo a questa Assemblea che solo nel Regno Unito sono stati depositati oltre 2.500.000 profili del DNA,

Questo Trattato, come ho già detto, giunge al termine di un complesso procedimento legislativo: l'adesione della Repubblica italiana era stata firmata il 27 maggio 2005 e inspiegabilmente per due anni, nella XV legislatura, non vi era stato il tempo tempo di portarlo ad esecuzione e alla ratifica del Presidente della Repubblica. Oggi, nonostante alcuni aspetti negativi sui trattamenti e sui finanziamenti per quanto riguarda il complesso sistema della sicurezza, che sono stati evocati dagli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto, possiamo mettere un segno positivo all'azione di Governo su questo tema credo che in questa direzione debbano essere anche rimeditati gli interventi e le rivendicazioni che gli organismi di rappresentanza dei corpi di Polizia militare (i COCER), e i sindacati di Polizia avevano più volte indirizzato all'azione di Governo e alla politica. Oggi, quindi, è davvero una giornata importante e dopo le scoperte che portarono nel secolo scorso all'identificazione dattiloscopica, finalmente possiamo utilizzare un altro strumento dell'evoluzione tecnico-scientifica per il contrasto ad ogni forma di criminalità. Da questo provvedimento naturalmente discende la conseguenza che occorrerà poi affrontare il tema dei trattamenti e dell'accertamento obbligatorio, che io reputo necessario per alcuni tipi di illeciti in materia ad esempio di reati commessi sotto l'effetto e l'intossicazione di sostanze alcoliche, e credo che lo strumento che utilizziamo per i prelievi ematici e per i prelievi attraverso cui si riesce ad operare l'identificazione del DNA potrà essere lo stesso strumento per l'accertamento di quei reati.

potremo finalmente frenare pericolosissimi fenomeni criminali che offendono la dignità della nostra società come gli omicidi e soprattutto le stragi, che in questo Paese hanno caratterizzato decenni

un accordo di carattere internazionale, è evidente che l'impianto non può che risentire di una certa uniformità ai principi ispiratori del Trattato.

da quelli che hanno caratterizzato l'azione del precedente Governo, che non è giunto all'approvazione del provvedimento medesimo. Voglio tra l'altro ricordare come l'impianto del provvedimento che oggi è sottoposto all'esame dell'Aula è frutto di un lavoro particolarmente approfondito, svolto con il concorso di tutti i componenti (prima del Comitato ristretto e poi delle Commissioni riunite nel loro *plenum*), che ha portato - ben ha fatto il collega Mazzatorta a ricordarlo - ad un'ottimizzazione dell'impianto affinché si avesse un particolare riguardo al profilo delle garanzie, avendo realizzato da questo punto di vista un un prodotto finito di altissimo livello tale da garantire che sotto questo aspetto non vi possano essere rilievi ed eccezioni di sorta. Con queste premesse, credo che si possa guardare all'approvazione di questo provvedimento

infatti, di politica di allocazione di risorse, che si presta sempre a valutazioni diverse sulle scelte opinabili e contrapponibili; parliamo di interessi del nostro Paese e questi normalmente - come accade anche in questa occasione - sono sempre auspicatamente ampiamente condivisi.

il correlatore Mugnai. Innanzitutto i cinque testi erano estremamente sovrapponibili, ma anche il testo presentato dal Governo, trattandosi del recepimento di una norma di diritto internazionale, non poteva che essere di natura pressoché identica. Se il senatore Li Gotti fosse stato attento nella relazione avevo esattamente citato che tutti i testi, compreso quello governativo, prendono origine dall'atto Senato n. 1877, presentato dal Governo Prodi e dai Ministri competenti di quel Governo. Noi possiamo dire,

Possiamo vedere sempre più forze di polizia che cooperano scambiandosi dati e notizie utili. Finalmente possono addirittura sconfinare per prevenire reati sul territorio di uno Stato

sui voli di linea non farà che rendere più sicuri i voli da ogni tipo di condotta che possa pregiudicare la sicurezza del volo. Sappiamo quanto oggi si faccia e quanto si possano temere

conto il dotarsi di una banca dati dei DNA, ossia avere la certezza delle identificazioni personali e il fatto di poter riscontrare, quando questa sarà attuata, una corrispondenza tra la persona che ha commesso un reato e dei campioni che si potranno rintracciare sui luoghi

si dovrà bloccare in questa fase, dovendo aspettare almeno una comunicazione del Ministero delle finanze, o se il Governo abbia già la soluzione o un emendamento da presentare in corso d'opera. In tal caso potremo dare il via immediato al recepimento del Trattato.

relatori, dai loro Presidenti, dal presidente Dini e soprattutto dal Comitato ristretto. Per il Governo l'approvazione del provvedimento in esame rappresenta la conferma del carattere prioritario della questione sicurezza.

svolgendo nelle Commissioni 1ª e 2ª riunite, attraverso il varo di due decreti legislativi in materia di ricongiungimenti familiari e di disciplina dell'asilo e, non da ultimo in termini di importanza, attraverso la ratifica del Trattato di Prum.

di persone la cui identità non sia certa e, soprattutto, di persone scomparse, tasto su cui vi è una sensibilità diffusa. Ricordo che esiste all'interno del Governo anche un commissario straordinario che ha il compito specifico di coordinare le iniziative tese al loro ritrovamento. Già i relatori hanno risposto a qualche intervento da parte di esponenti dell'opposizione

la Commissione parlamentare antimafia aveva elaborato proposte molto interessanti, così come il Governo della passata legislatura elaborato dei disegni di legge che contenevano in materia di sicurezza passaggi molto interessanti. In questa legislatura stiamo traducendo i suddetti passaggi in norme concrete ed operative. Ciò significa che questo Governo e la maggioranza che lo sostiene non valutano queste tematiche sulla base del colore di chi le ha elaborate, ma sulla base della loro oggettiva validità, e significa altresì che hanno la forza politica per approvarle. Forse è questo che segna la differenza rispetto al passato.

L'auspicio del Governo è che questo possa avvenire prima della pausa delle festività natalizie, in modo tale da permettere nei tempi più rapidi all'altro ramo del Parlamento di varare definitivamente questo importante Trattato.

Signor Presidente, vorrei che fosse verbalizzata la mia partecipazione all'ultima votazione relativamente all'approvazione del disegno di legge n. 1152-B, che per qualche disguido della mia postazione telematica non è stata registrata. Nel mentre ho fatto il controllo era già iniziata la discussione sul provvedimento; non ho chiesto subito la parola ma ho fatto rilevare agli Uffici preposti

card*. Abbiamo sentito il Governo promettere per bocca di Giulio Tremonti quanto segue: «Il buon avvio rende giustizia di tante ironie che si erano sentite. La carta sarà caricata entro due giorni lavorativi».

da una settimana e quando provano a ritirare i soldi la carta risulta scarica. Sempre sui quotidiani leggo una dichiarazione del Ministero dell'economia che dice: che dice: «Conosciamo il problema, ma abbiamo ricevuto troppe richieste. Non ce lo aspettavamo». Non è possibile scherzare con persone che hanno un reddito inferiore a 6.000 euro l'anno

sulle pensioni e sui salari. Invece, si è voluto fare un'operazione di propaganda con la *card*, che tra l'altro serve anche per le ricariche degli operatori. Ma lasciamo stare, dato che non è questa la sede per dare giudizi

una nuova finestra"). La Presidenza verificherà e solleciterà il Governo sulla possibilità di un'informativa urgente nei termini che lei ha chiesto. Lei stessa forse può fare anche un'interrogazione